I Presidenti del Senato e della Camera dei deputati hanno proceduto alla nomina dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, il cui elenco è pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna. La Commissione, convocata oggi alle ore 13, ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza. Sono risultati eletti: Presidente: deputato Jacopo Morrone; Vice Presidenti: deputati Gerolamo Cangiano e Francesco Emilio Borrelli; Segretari: deputati Dario Iaia e Marco Simiani. Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e di vigilanza in materia di immigrazione, convocato oggi alle ore 14, ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

e della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. L'elenco dei componenti delle due Commissioni è pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna. Le Commissioni sono convocate per la loro costituzione domani, mercoledì 13 settembre, nella sede di Palazzo San Macuto secondo i seguenti orari:

Signor Presidente, mi sembrava opportuno in questa sede - quindi la ringrazio per avermelo concesso - ricordare il professor De Masi. Questo significa rendergli l'omaggio che merita. In qualità di intellettuale del nostro Paese ha contribuito in modo scientifico e puntuale, con la vivacità tipica di chi è gioioso e intelligente, ad arricchire il dibattito pubblico sui temi che vedono la politica e la società come protagoniste. In realtà, gli farei un grave torto se oggi qui svilissi il suo pensiero, provando a riassumerlo. Non basterebbero i minuti - sicuramente pochi - a disposizione per sintetizzare i temi che ha studiato con scientifica dedizione, con anni e anni di duro lavoro di ricerca. Sono e saranno le sue innumerevoli pubblicazioni scientifiche, i libri divulgativi, gli importanti e autorevoli incarichi e ruoli universitari e i contributi alle strutture organizzative pubbliche e private, a ricordarci l'eredità che oggi tutti possiamo raccogliere. Dico tutti perché le idee del professor De Masi, seppur ideologicamente definite e chiare, non servono solo a chi le sposa e le condivide, ma anche - forse soprattutto - servono a chi ha l'arduo compito di controbatterle per destrutturarle, argomentando. Del resto è a questo che servono gli intellettuali. Del professor De Masi parleranno in ogni luogo anche molti *manager*, professori e professionisti che hanno avuto l'onore di essere formati da lui. Del valore della sua umanità e personalità sono testimoni illustri amici e intellettuali di cui si circondava, dal presidente del Brasile, Lula, a personalità come Sciascia, Pasolini ed altri. ed altri. Il professor De Masi credeva fortemente nel metodo scientifico e quindi all'incrocio dei dati e alla consequenzialità degli stessi rispetto alle idee e spesso mi diceva che in questo suo nuovo ruolo non sopportava che in TV lo intervistassero insieme a degli opinionisti, perché non va bene che chi ha studiato tanto una materia debba dibattere con chi quella materia non l'ha studiata. Oggi, però, vorrei ricordarlo non dal punto di vista intellettuale, ma dal punto di vista Sapete bene che spesso gli è stato dato, svilendolo, del grillino, non certo svilendo la storia del MoVimento, ma certamente per noi è stato un riferimento. Mi dispiace ricordarlo con questo brusìo, perché credo che la politica tutta, di destra e di sinistra, abbia bisogno di intellettuali anche quando di questi non si condividono le idee. È proprio dalle ricerche e dalla loro sintesi che forse dovremmo riuscire a costruire un dibattito più maturo e meno tipico dei *talk show*. Con noi ha condotto diverse ricerche, dal lavoro alla cultura, non ultima quella fatta con me sul MoVimento stesso. C'è una sua semplicissima frase che mi piace ricordare. Quando gli chiesi di aiutarmi a portare avanti un'indagine sulla natura stessa del MoVimento in piena pandemia, mi disse che era meraviglioso che una forza politica si facesse delle domande e si chiedesse quale tipo di società vorremmo per il futuro e mi ricordava sempre che il futuro non si aspetta: il futuro prima bisogna fare la fatica di immaginarlo e dopo la fatica ancora maggiore di provare a costruirlo e non contro tutti e tutto, ma con tutti e con tutto. Per noi è una grave perdita, personalmente mi permetterete, in conclusione, di confidarvi alcuni ricordi di Mimmo (da adesso avrei piacere di chiamarlo così). Ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo sempre di più, mi ha concesso con naturale semplicità e con mia meraviglia la sua amicizia e a volte mi sono chiesta perché trascorresse del tempo con me, progettando scuole, idee, eventi e pensavo di essere come un topo di laboratorio. Ho pensato persino che mi stesse studiando da sociologo per capire come erano fatti questi grillini visti da vicino, ma poi vedevo i suoi occhi, il piacere del nostro incontro e percepivo una stima che ho avuto - credetemi - l'ardire e persino la boria di raccogliere tutta di tenere stretta a me, pensandomi migliore solo perché lui mi stimava e questo mi ha spronata ad essere migliore per meritarla. Mi sono presa l'amicizia così come è nata. Una sola curiosità: sapete cosa diceva spesso a me e agli amici? Mi chiedeva: Barbara, ma sei felice? Riesci a prendere del tempo per te? Sì, perché lui si preoccupava della felicità e del tempo. Ecco il grande insegnamento politico che ci lascia: la felicità e il tempo devono diventare temi politici, mi ha detto. È la politica che deve restituire alle persone il tempo e deve dare loro gli strumenti perché esse siano felici. Non abbiate timore di parlare di questi temi in Parlamento, ce n'è un gran bisogno ed è il vero nuovo lusso. Mi diceva: se non combatterete le ingiustizie sociali che impediscono alle persone di essere felici e di avere tempo, Barbara, anche voi grillini avrete fallito. Mimmo è morto a ottantacinque anni ed era il più giovane di noi; è volato via, come diceva lui, leggero come una rondine ma non come una piuma, perché una rondine sa bene dove vuole andare. Il MoVimento ha perso un intellettuale di riferimento, io ho perso un maestro e un amico. Senatrice Floridia, penso che la scomparsa del professor De Masi non sia solamente una perdita per il MoVimento 5 Stelle, ma per tutto il Paese. Penso quindi che sia giusto che il Senato gli dedichi un minuto di riflessione. *(Il

Presidente

ricordo di Mimmo De Masi, che non è stato solo un grande accademico, un sociologo raffinato e un intellettuale apprezzato da tutti. È stato un uomo libero, un uomo che ha detto sempre la sua, spesso controvento, tantissime volte controcorrente, quasi sempre però interpretando i i cambiamenti sociali che accompagnavano le grandi trasformazioni. A Mimmo De Masi ci legherà sempre il rapporto schietto che ha avuto con la nostra comunità e con tante e tanti di noi, anche nei momenti più complicati e più difficili della storia recente del nostro Paese. Ci auguriamo, come proporremo in una delle prossime riunioni della Conferenza dei Presidenti, che si possa riflettere su molti suoi scritti in un momento dedicato, *ad hoc*, magari davanti anche alla sua famiglia, che ieri abbiamo salutato tutti con grande affetto. Ho chiesto la parola, signor Presidente, per sottoporre all'attenzione dell'Assemblea alcune difficoltà oggettive - mi rivolgo al sottosegretario Bitonci e, attraverso lui, al resto del Governo - perché troviamo oggettivamente inaccettabile che anche alla riapertura dei lavori si riprenda con le vecchie pratiche. Ci eravamo assicurati reciprocamente, non dico un *time out*, sottosegretario Bitonci, ma almeno un confronto preventivo sul modello dei nostri lavori. Richiamo l'attenzione dell'Assemblea non solo sul contenuto

è che nella XIX legislatura, dopo appena dieci mesi dall'insediamento del Governo, sono stati già emanati 38 decreti-legge, a cui si aggiungono tre decreti-legge approvati dal Consiglio dei ministri, in attesa di pubblicazione (non sappiamo quando vedremo i testi). Nei

di un atto generico nel merito e nelle coperture finanziarie. La cosa che ci preoccupa - lo dico ai colleghi di tutti i Gruppi parlamentari - è che stiamo autorizzando una spesa da 2,5 miliardi chiudendo gli occhi,

le preleviamo dal patrimonio destinato - ricordo a tutti noi che il Governo era stato autorizzato ad emettere titoli per 44 miliardi - ma ad oggi non sappiamo né quanti titoli sono stati emessi, né a quanto ammonta il fondo,

in 8a e in 9a Commissione hanno già contestato il fatto che fosse confluito un decreto intero dentro un altro provvedimento, che è un *omnibus*. Signor Presidente, dobbiamo capirci: se ricominciamo così, non so dove andremo a finire in sede di legge di bilancio. Vorrei che questo aspetto non riguardasse solo l'opposizione, perché la modalità con cui legiferiamo riguarda tutti noi. Eravamo stati rassicurati, quando ci siamo salutati prima della

cosiddetto TIM che confluisce in un decreto *omnibus*. Lo diciamo senza giri di parole: chiediamo al Governo il ritiro dell'emendamento TIM dal decreto *omnibus*, l'esame approfondito nelle Commissioni di merito di quel decreto e la produzione di una relazione tecnica dettagliata sul provvedimento. Ci aspettiamo che il MEF ci dica dove vanno quelle risorse e che il Ministero dello sviluppo economico batta un colpo, perché di politiche industriali e di politiche connesse al futuro dei lavoratori di quel comparto non c'è traccia. Signor Presidente, vorrei fare presente che, nell'ultima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, il ministro Ciriani aveva annunciato l'intenzione da parte del Governo di il decreto-legge cosiddetto TIM in un altro decreto. Come lo stesso presidente Boccia ha ricordato, non è una novità: l'abbiamo visto accadere parecchie volte nel passato.

procedere nel modo più ordinato possibile per quanto riguarda la legislazione, ma devo dire che se c'è stato un alto numero di decreti è perché c'è stata un'attività è perché c'è stata un'attività legislativa molto intensa che ha introdotto una serie di misure, che stanno tra l'altro mostrando i loro effetti, come dicono i

confluenza è stata annunciata dal ministro Ciriani in Conferenza dei Capigruppo, senza che venissero sollevate obiezioni.

la relazione. Per quanto riguarda i contenuti, rinvio alla relazione che accompagna il provvedimento. Essendo, però, un disegno di legge delega, che avrà quindi un seguito, credo sia giusto sottolineare giusto sottolineare ulteriormente come il lavoro in Commissione, anche da parte del Governo, con il sottosegretario Bitonci, sia stato davvero particolarmente costruttivo condiviso tra maggioranza e opposizione. Come metodo di lavoro, abbiamo adottato una condivisione, che, lo ripeto, è stata costruttiva, che ha portato anche a riformulare emendamenti, individuando elementi comuni da parte di tutti i Gruppi. D'altra parte, l'argomento si presta alla possibilità di ricostruire un sistema di incentivi finanziari alle imprese che non ci faccia perdere risorse e che possa individuare gli ambiti nei quali il nostro sistema produttivo e industriale possa davvero ritornare a correre, come tutti ci auguriamo. questi elementi comuni, ritrovati fra tutti i Gruppi, hanno portato a una conseguente approvazione di testi concordati e identici tra loro.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il bisogno è noto. Lo riporta la relazione illustrativa, lo hanno riferito diversi auditi emerso nei lavori della Commissione. È chiaro a chiunque di noi dialoghi con imprenditori e aziende, che il sistema degli incentivi alle imprese ha bisogno di organicità e di coerenza. Vedete, colleghi, come in altri settori di politica pubblica, anche in materia di sovvenzioni il nostro Paese sconta un sistema eterogeneo, costruito su stratificazioni successive, sovrapposizioni di linee di politica nazionale, prassi regionali e l'adozione di principi, procedure e strumenti mutuati dalla programmazione comunitaria, che sono diventati regola per la spesa dei fondi strutturali e poi prassi, anche nella programmazione con fondi nazionali. In questo contesto, è sicuramente necessario che questo corpo di stratificazioni successive acquisisca un ordine, una struttura organica e diventi appunto un sistema di incentivi. Questo provvedimento va nella giusta direzione. Si mira a definire gli obiettivi e i principi che tale disciplina organica dovrà avere e a definire il perimetro della delega. Ma l'organicità delle procedure è solo uno dei bisogni di fondo. abbiamo anche la forte necessità di strumenti per misurare e valutare l'impatto degli interventi. Capacità di misurazione e valutazione degli impatti sono un'esigenza strategica per le politiche pubbliche di investimento su cui il nostro Paese ha tanto da lavorare. Ancora, dotarsi di un organismo di valutazione, di infrastrutture digitali interoperabili in grado di coadiuvare le imprese, di strumenti per determinare l'impatto: questi sono temi che il futuro sistema delle sovvenzioni alle imprese deve definire e sono contenuti tra i principi enunciati nel provvedimento che oggi andiamo ad analizzare. Quindi, condividiamo la finalità e l'ambito di applicazione del disegno di legge in esame. Come MoVimento 5 Stelle, abbiamo già dimostrato di non avere pregiudizi politici nel supportare interventi che mirano a sostenere il sistema produttivo e di certo non li avremo oggi, su questo provvedimento. il provvedimento in cui maggiormente c'è stato confronto, coordinamento e capacità di sintesi tra le forze politiche di opposizione e di maggioranza. Al riguardo vorrei ringraziare tutti i componenti della 9a Commissione, il presidente De Carlo e il senatore Paroli, con i quali è stato possibile intavolare un confronto

spirito di cooperazione nella stesura del decreto legislativo che darà corpo e sostanza ai principi che stiamo definendo oggi, perché sarà questo a determinare il reale impatto del sistema di incentivi. C'è da scongiurare che i principi, che necessariamente sotto certi aspetti sono ampi, non del tutto circoscritti o definiti, si possano tradurre in una delega in bianco. Speriamo di no.

intanto proprio dal passaggio in 9a Commissione, nell'articolo 1, che circoscrive l'ambito della delega e ne stabilisce le finalità, è stato opportunamente inserito un richiamo esplicito all'articolo 117 della Costituzione. Deve essere chiaro - e dovrà esserlo anche nella scelta degli strumenti e delle procedure - che tra gli obiettivi del sistema delle sovvenzioni deve deve esserci la riduzione del divario socioeconomico tra Nord e Sud. Questo non è un richiamo scontato se si pensa che attualmente il Nord ottiene l'86 per cento degli incentivi e che in passato per parte della politica è stata pacifica una sorta di ripartizione funzionale delle risorse per lo sviluppo: sovvenzioni alle imprese del Nord, aiuti agli investimenti strutturali al Sud. La coesione territoriale passa dalle infrastrutture, ma anche dal rafforzamento del tessuto produttivo. Non ci serve un ponte sullo Stretto; al Sud servono certamente le infrastrutture, ma serve anche e soprattutto che sullo Stretto, sulla tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, sui porti sardi le merci viaggino in entrambe le direzioni e non quasi esclusivamente da Nord verso Sud. *(Applausi)*. Per far questo dobbiamo far crescere il tessuto delle imprese del Sud, anche agendo su un sistema di sovvenzioni che sia basato sui principi di piena coesione territoriale e quindi sui principi dell'articolo 117 della Costituzione. È stato esteso l'ambito delle sovvenzioni agli incentivi fiscali. Considerare le sovvenzioni in maniera complessiva a prescindere dalla leva che utilizzano (quindi fiscale, conto capitale, eccetera) è la prima chiave per rendere organico il sistema e costituire una specifica disciplina di settore. Tra i principi sono richiamati esplicitamente la pluriennalità e la certezza dell'orizzonte temporale, principio cardine per le imprese che hanno bisogno di un quadro stabile, certo e affidabile delle politiche di incentivo. Peccato non lo abbiate previsto prima, perché magari vi avrebbe dissuaso dal devastare una misura di grande impatto come il superbonus 110 per cento senza nessuna strategia, senza nessun principio se non quello di distruggere il lavoro del MoVimento 5 Stelle per contrasto politico, mandando in confusione un intero settore e mettendo in ginocchio migliaia di imprese. Non sono io a

Paese. In chiusura vorrei soffermarmi su due principi fondamentali correlati: quello dell'agevole conoscibilità delle misure da parte degli imprenditori e della digitalizzazione delle procedure. Su questo fronte ci aspettiamo non soltanto portali per la diffusione delle informazioni, ma una reale valorizzazione degli *open data* in possesso della nostra pubblica amministrazione, a partire dalle banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, che permettano alle amministrazioni di fare analisi sugli impatti delle politiche di aiuto e alle imprese di capire e valutare la dimensione e le caratteristiche delle misure disponibili. la digitalizzazione delle procedure, per essere equa, deve passare da una digitalizzazione del Paese. In attesa di un accesso uniforme alla banda larga, procedure come il *click day* sono discriminatorie per le imprese insediate in alcune aree del Paese. Per questo avremmo gradito un'esplicita esclusione del *click day* e come MoVimento 5 Stelle avevamo proposto un emendamento in tal senso. La riformulazione non ci lascia pienamente soddisfatti e infatti ci riproveremo. Nel complesso, comunque, la delega incontra il nostro favore, così come il metodo e il clima di lavoro che hanno portato alla sua definizione. Ora speriamo, ci aspettiamo, consideriamo imprescindibile che la stessa collaborazione si abbia nel definire il sistema degli a livello internazionale, riveste un'importanza strategica per il futuro del nostro Paese. Ricordiamoci che nel 2021 l'ammontare delle agevolazioni complessivamente concesse, per quanto riguarda il tema degli incentivi diretti alle imprese (agevolazioni fiscali, crediti d'imposta, interventi a garanzia e sgravi contributivi), ha raggiunto la cifra di 146 miliardi di euro. In particolare, gli incentivi diretti alle imprese sono stati in tutto 25 miliardi. Escludendo gli interventi gestiti dall'Agenzia delle entrate (gli interventi a garanzia), nel 2021 le amministrazioni centrali e regionali hanno approvato quasi 700.000 domande alle aziende. Nel complesso, gli investimenti attivati a sostegno di tali incentivi sono stati pari a 314 miliardi di euro: un volano economico straordinario, con un rilevante impatto sull'economia italiana. Nel corso dell'esame del disegno di legge delega sugli incentivi,

il Governo e il sottosegretario Bitonci per l'impegno profuso. Più volte in Commissione abbiamo discusso, affrontato e limato; alla fine è uscito un testo che ha ottenuto il massimo consenso possibile nell'ambito della Commissione (ognuno nelle proprie vesti). L'importante abbiamo dato dei contributi forti al Governo per quanto riguarda la delega su questo tema, inserendo alcune novità e allargando agli aiuti fiscali, con l'inclusione del bonus 5.0. Nel merito, viene peraltro potenziato il coordinamento con le Regioni; si chiarisce che la revisione includerà gli incentivi alle imprese di natura fiscale; viene fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e controllo, demandata, questa, a una specifica disciplina di settore, settore, in modo da poter intervenire, con i successivi decreti delegati, anche sul tema dei crediti di imposta del Piano transizione 4.0 gestiti dal Mimit. Sono stati inseriti poi gli emendamenti che recepiscono le preoccupazioni sollevate dalle Regioni sul rischio di una razionalizzazione, con relativo taglio delle misure, decisa direttamente dal Ministero. Di qui l'approvazione di correttivi che richiamano al rispetto delle competenze in materia, e soprattutto all'autonomia programmatica delle Regioni, anche sul cofinanziamento dei fondi europei, e sanciscono l'autonomia nell'individuazione di eventuali modelli di riordino e nell'attuazione di specifici interventi mirati, comunque nel rispetto delle diverse realtà territoriali. Ritengo comunque che si dovrà lavorare ancora sul tema del *click day*, che in molti casi trasforma l'accesso delle imprese agli incentivi in una corsa *online*. In questo caso è stato inserito un riferimento all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali, che riducano il rischio che l'assegnazione avvenga sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza. Tra i vari emendamenti approvati, cito quello a firma del nostro movimento, che riveste particolare importanza e inserisce tra i destinatari degli incentivi anche i professionisti, introducendo il principio che la qualificazione di professionista non è di ostacolo alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti, ove ne ricorrano i presupposti. A questo proposito, ricordo che si tratta di una riformulazione di un emendamento che sanciva il principio di piena equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361 - ogni tanto qualcosa di buono lo fa - che considera impresa qualsiasi entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita, incluse in particolare le entità che svolgono attività artigianali, attività a titolo individuale o familiare, le società di persone e le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica. Altre novità riguardano gli incentivi di natura fiscale. Con un altro emendamento si prevede infatti che la revisione delle misure agevolative deve includere altresì gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, mentre gli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo degli incentivi stessi sono demandati alla specifica disciplina di settore, ossia alla delega fiscale. In base alla formulazione che esce dalla nostra Commissione, pertanto, il processo di revisione deve puntare alla sistematizzazione degli strumenti agevolativi esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti e/o delle finalità dell'agevolazione, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione, all'innovazione, alla sostenibilità ambientale, nonché alla facilitazione nell'accesso al credito delle imprese, al rafforzamento patrimoniale delle stesse, alla crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione o altri ambiti e finalità di sostegno. Ricordo, infine, che particolare attenzione è stata attribuita ai requisiti premianti, riservando specifica considerazione, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, oltreché al lavoro e alle imprese femminili, anche e soprattutto al lavoro giovanile. complessivamente per il ruolo che ricopriamo abbiamo il dovere di sostenere con tutti i mezzi a nostra disposizione i nostri imprenditori, creando il migliore contesto competitivo per poterli agevolare, permettendo loro di competere a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale, ricordando quanto diceva Keynes, ovvero investire con successo significa anticipare le anticipazioni degli altri. *(Applausi)*. il disegno di legge delega che riscrive il complesso sistema degli incentivi alle imprese ha avuto un lungo e articolato esame nella Commissione del Senato che si occupa di attività produttive. Sono state decine le audizioni degli *stakeholder*, cioè le imprese, le confederazioni, gli enti e le istituzioni che hanno voluto dare il proprio contributo per dedicarsi al complesso insieme di incentivi vigenti. Essi hanno anche suggerito idee, punti di vista e soluzioni per ridisegnare il nuovo sistema di sostegni pubblici. Tutti hanno voluto portare il proprio contributo fattivo e ragionato in una delega che, essendo stata scritta dal Governo, aveva già avuto un'impronta e un confronto a più alti livelli. La 9a Commissione, grazie a un ascolto molto attento da parte del relatore Paroli e del sottosegretario Bitonci, ha voluto ulteriormente migliorare il testo, accogliendo le proposte emendative provenienti anche dalle opposizioni. Si è arrivati, quindi, a un testo largamente condiviso, che lascia al lavoro di decreti delegati la definizione finale del quadro di aiuti, incentivi e contributi: un insieme di norme che dovrà tenere conto anche della necessità - pure condivisa in Commissione - di arrivare a una semplificazione delle procedure e alla produzione di documentazione per i richiedenti gli incentivi. L'altro tema che risulta evidente dalla delega è che si dovrà evitare quel vasto spreco di risorse che spesso non raggiungono gli scopi per cui sono state concepite. Questo purtroppo spesso avviene nel Mezzogiorno ed è uno dei motivi della mancata crescita di alcuni territori. Gli incentivi, pertanto, devono avere una finalizzazione precisa e devono andare a progetti che abbiano un impatto evidente anche sull'economia dei territori in cui arrivano. L'altro tema affrontato è quello della semplificazione delle procedure e della certezza del procedimento finalizzato a concedere gli incentivi. Le domande dovranno essere presentate attraverso procedure semplici e oggettive, evitando l'accesso a misure la cui selezione sia lasciata solo a chi arriva La previsione di un portale unico degli incentivi pubblici, oggi parcellatizzati in oltre 1.900 diverse misure, potrà aiutare gli imprenditori alla ricerca dell'incentivo più adatto alla propria impresa. Gli obiettivi sono la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese per aiutarle a competere sui mercati, anche su quelli globali, posto che la gran parte delle nostre imprese ha ancora dimensione ridotte per competere a livello internazionale.

Quindi, se è vero che i decreti delegati dovranno vedere la luce entro due anni dall'approvazione definitiva della delega, verosimilmente entro la seconda metà del 2025, è altrettanto vero che i finanziamenti del PNRR dovranno operare con la stessa logica prevista da questa delega. La revisione del Piano, che abbiamo letto e discusso ai primi di agosto, va nella direzione di razionalizzare gli interventi, di finanziare solo progetti realizzabili, di ottimizzare e non sprecare le risorse. Incentivi mirati, valutata la sostenibilità e la realizzazione dei progetti, sono la guida del complesso di norme che tiene insieme questa delega. La valutazione va fatta anche sul ritorno dell'investimento, cioè su quale sarà il suo impatto e quindi quale sarà il moltiplicatore dell'incentivo pubblico. Il tema è non sprecare risorse per incentivi che abbiano un impatto limitato, addirittura inferiore al valore dell'incentivo, come spesso è successo. C'è quindi il tema del coordinamento tra gli incentivi delle amministrazioni pubbliche statali e quelle delle amministrazioni del territorio, che dovranno non sovrapporsi, ma ottenere ma ottenere il miglior risultato ove sia prevista una compartecipazione tra incentivi statali e regionali. Per definire un quadro organico di incentivo è prevista anche la redazione di un apposito codice degli incentivi, che dovrà contenere e armonizzare tutta la disciplina in materia. La delega prevede il rispetto di principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nella scrittura del codice. L'altro principio guida è quello di sistematizzare le risorse a disposizione degli incentivi, tenuto conto della normativa europea, *in primis* il Trattato sull'Unione, che ha criteri molto rigidi per definire l'ammissibilità degli aiuti e la loro incompatibilità con gli aiuti di Stato. vanno inquadrate e programmate *a priori*, senza incorrere in eventuali bocciature della Commissione europea. La programmazione deve essere pluriennale, osservare precisi obiettivi strategici di sviluppo con tipologie prestabilite, con un cronoprogramma relativo all'attuazione degli interventi e alla definizione del quadro finanziario delle risorse necessarie alla realizzazione di progetti. Un'attenzione particolare dovrà essere riservata agli incentivi mirati a valorizzare il lavoro femminile, quello dei giovani e dei disabili. Come abbiamo detto, la semplificazione delle procedure è l'altro punto qualificante di questa delega, per cui da parte delle amministrazioni concedenti gli incentivi dovranno essere previsti il rispetto dei tempi delle attività istruttorie, la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi. In questo quadro rientrano la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure anche in materia di controlli. Gli interventi e la loro efficacia verranno valutati in tutte le fasi di realizzazione, da quella progettuale a quella esecutiva, a quella finale. Importante è la svolta verso la sburocratizzazione, la modernizzazione e la digitalizzazione Vorrei ricordare che diversi sono gli emendamenti di Forza Italia che sono stati accolti durante l'esame in Commissione, dove il lavoro è stato corale e fattivo. Tutti i Gruppi hanno trovato ascolto sulle proprie proposte emendative da parte del relatore e del Governo. Insomma, si tratta di un provvedimento che finalmente crea un quadro di regole per una delega in materia di incentivi alle imprese largamente condivisa dai diversi schieramenti politici e che vede Forza Italia assolutamente favorevole. Presidente, Sottosegretario, colleghi, stiamo discutendo di un disegno di legge delega che mira ad adottare entro due anni uno o più decreti legislativi che definiscano un quadro organico degli incentivi utili a sostenere le imprese nelle forme più idonee ed efficaci possibili. Ci si aspetta un sostegno del tessuto produttivo mediante un'indispensabile pianificazione. Dunque, è una revisione del sistema di incentivi alle imprese e di semplificazione delle relative procedure. La programmazione di interventi dovrebbe avvenire in modo da assicurare un sostegno continuativo e pluriennale. È importante che sia in raccordo con il sistema degli incentivi regionali e quelli finanziati dai fondi europei, appunto per evitare sovrapposizioni. È un disegno di legge che rappresenta senza dubbio un'occasione per fare il punto e soprattutto stabilire soluzioni normative su una serie di tematiche scottanti, che continuano ad affliggere il sistema economico nazionale. Parto da quella per me più grave e decisamente ingiustificabile: la tematica relativa al Mezzogiorno e alla crescita a due velocità che distanzia il Nord dal Sud. Da questo punto di vista, la politica degli incentivi alle imprese deve cambiare rotta e dare una sferzata di vitalità al tessuto economico del Paese nella sua interezza. Purtroppo, invece, appare ancora allocata in una misura disomogenea a svantaggio del Meridione, che vede troppe mancate occasioni, diretta causa della carenza occupazionale e dunque di emigrazione e spopolamento di ormai davvero troppi centri urbani. È chiaro ormai che, soprattutto per le aree svantaggiate, occorre investire e occorre farlo per la valorizzazione delle eccellenze presenti sui territori. È un dovere agevolarle in difesa del nostro *made in Italy*, supportando le progettualità e la ricerca, facilitando il trasferimento tecnologico, sostenendo il capitale umano, continuando a far sì che vi siano la circolazione e la condivisione delle conoscenze, anche con l'ausilio di strutturati corsi di formazione tanto auspicati. Viviamo un contesto industriale - e non solo - in continuo mutamento. Dunque, è necessario avvalersi di circuiti innovativi e resilienti in grado di rispondere in maniera flessibile al costante cambiamento dei modelli produttivi e così incidere positivamente sulla crescita economica nazionale. Questo disegno di legge delega inserisce tra gli obiettivi l'individuazione di un insieme definito di modelli agevolativi selezionati in base ai risultati riscontrati. C'è da dire che è un ottimo proposito per mettere in campo ausili utili e funzionali all'attività di impresa. Altro importante tema che abbiamo affrontato nel lavoro emendativo in Commissione riguarda un buon 50 per cento della popolazione, vale a dire la questione della disparità di genere. Secondo il *report* di Unioncamere sull'imprenditoria femminile dello scorso luglio, in Italia le imprese femminili sono più di 1,3 milioni, su un totale di 6 milioni. Si tratta per lo più di microimprese e piccole imprese. Soltanto lo 0,3 per cento delle imprese di medie o grandi dimensioni è guidato da donne. Quest'ultimo dato è solo uno dei tanti sintomi del forte ritardo che l'Italia sconta in termini di parità di genere. Le altre spie di allarme di questo malessere socio-economico sono la bassa occupazione, un inaccettabile differenziale salariale pari a circa il 20 per cento in meno rispetto agli uomini e forme contrattuali penalizzanti. Le donne - come se non bastasse - hanno pagato il prezzo più caro durante l'emergenza sanitaria: persi su quattro nel primo anno della pandemia e questo dato può estendersi, purtroppo, anche all'occupazione giovanile. La ripresa non è stata delle migliori, con forme di contrattualizzazione a singhiozzo che non hanno fatto altro che aumentare le differenze, evidenziando più che mai la necessità di concreti servizi di *welfare* aziendale che generino stabilità e imprimano una visione strutturale, servizi utili a sviluppare sinergie virtuose e complementari con il sistema del *welfare* pubblico, specialmente in momenti delicati come quello della maternità e del ritorno a seguito della maternità, certamente più complesso sotto il profilo della gestione dei nuovi equilibri che inevitabilmente si vengono a creare. Un altro aspetto su cui, con il mio Gruppo, abbiamo ritenuto fondamentale accendere un faro è quello relativo alla previsione di premialità per le imprese che svolgono attività ecosostenibili e a basso impatto ambientale. Ancora una volta, quindi, proprio nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, non si può e non si deve più prescindere da questo tema perché si collega a doppio filo con i drammatici impatti funesti del cambiamento climatico. Più imprese saranno incoraggiate e maggiori saranno gli effetti positivi sul piano ambientale, in un circuito verde sempre più rispettoso delle risorse del pianeta. La parte più attesa, cioè quella che riguarda gli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo degli incentivi aventi natura fiscale, è demandata alla specifica disciplina di settore, cioè alla delega fiscale. L'impegno e l'attenzione dunque continueranno senza sosta al fianco dei cittadini e per i cittadini, affinché il fare impresa diventi un volano sicuro per l'economia italiana tutta. *(Applausi)*.

Il provvedimento nasce dalla necessità di avere finalmente una riforma organica che metta ordine alla giungla degli incentivi, come chiesto a gran voce da tutte le associazioni di categoria. Il mondo produttivo italiano ha bisogno, oggi più che mai, di un sistema di incentivi ordinato e coordinato, che permetta alle imprese italiane di essere sempre più competitive per vincere le sfide globali che devono affrontare ogni giorno. Come emerge dalla relazione illustrativa, infatti, il quadro attuale degli incentivi appare molto confuso, con quasi 2.000 incentivi nazionali regionali spesso in contraddizione tra loro. Nel 2021, ad esempio, si sono registrati 1.982 interventi agevolativi, di cui 229 di natura nazionale e 1.753 di natura regionale, affidati alla gestione di 643 soggetti concedenti. Di fronte a un contesto così complesso e articolato, aggravato dal peso della burocrazia italiana, si comprende benissimo la richiesta da parte delle imprese di un intervento legislativo di riordino dell'intero sistema per assicurare una migliore pianificazione di tutti gli incentivi pubblici a sostegno del tessuto del tessuto produttivo. Il presente disegno di legge si muove proprio in questa direzione, riorganizzando in profondità il sistema degli incentivi affinché siano veramente in grado di stimolare investimenti innovativi e di garantire un supporto concreto in tutte le fasi di sviluppo dell'azienda. Entrando più nel dettaglio il disegno di legge incentivi introduce una serie di importanti novità e ha l'obiettivo di dotare il Paese di un sistema di strumenti fiscali e di selezione finanziaria chiari e semplici nella struttura e nelle modalità operative, con tempi di attuazione certi e con la possibilità di essere adattati a seconda delle diverse priorità e strategie che possono cambiare nel corso del tempo. In questo contesto vanno segnalati anche gli interventi per riportare gli incentivi nazionali e regionali all'interno di uno schema coerente e razionale, garantendo in questo modo il coordinamento tra le diverse misure, sempre però nel rispetto dell'autonomia regionale, come previsto dai nostri emendamenti. legge introduce anche la positiva novità del codice degli incentivi che punta a essere il testo di riferimento unico in materia di incentivi: un codice dotato di linee guida chiare che, tra le altre cose, ha il compito di semplificare le modalità operative e di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Un altro aspetto fondamentale contenuto nel provvedimento è la pianificazione pluriennale degli incentivi per assicurare alle imprese una prospettiva temporale certa di medio e lungo periodo. Questo è un elemento essenziale se vogliamo che la nostra industria possa competere con le industrie americana e cinese, le quali godono di investimenti spropositati rispetto alla realtà italiana ed europea. con una pianificazione di medio e lungo termine degli investimenti sarà possibile elaborare una serie politica industriale italiana e difendere veramente gli interessi nazionali. Il disegno di legge è stato positivamente arricchito e migliorato durante i lavori della Commissione. Tra i numerosi emendamenti e ordini del giorno proposti dalla Lega e approvati dalla Commissione, mi preme sottolineare l'emendamento che equipara i professionisti alle imprese e che consentirà quindi anche ai professionisti di beneficiare degli incentivi; un risultato storico che mette fine a una disparità di trattamento inaccettabile tra categorie e che garantisce finalmente pari opportunità a tutte le forze economiche che contribuiscono alla crescita del nostro Paese. un risultato questo importantissimo, atteso da migliaia di professionisti, per il quale ringraziamo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci. Ringrazio il Sottosegretario anche per la sua costante presenza in Commissione che ha agevolato il nostro lavoro e contribuito a migliorare il testo. Ancora una volta, anche con questo disegno di legge, la Lega e il Governo di centrodestra stanno dimostrando con i fatti di essere al lavoro per realizzare il programma elettorale che è stato premiato dal voto della maggioranza degli italiani. Noi siamo e saremo sempre dalla parte di chi lavora e di chi produce, dalla parte di chi crea lavoro e opportunità di crescita. Tagliare la burocrazia, abbattere le tasse, sostenere le imprese e le partite IVA, difendere il *made in Italy*, creare posti di lavoro: sono queste le priorità della nostra azione della nostra azione politica; sono queste le cose che stiamo facendo al Governo e che dobbiamo continuare a fare ogni giorno di più per far crescere il nostro Paese e per costruire un futuro di sviluppo e benessere per tutti gli italiani.

Noi riteniamo invece che rappresenti un tema centrale per la crescita del nostro Paese e che per questo dovrebbe trovare la massima attenzione della politica e delle istituzioni. Il sistema degli incentivi fornisce infatti in Italia, come nella maggior parte dei Paesi industrializzati, il principale strumento di qualsiasi progetto di politica industriale finalizzata a promuovere e facilitare l'innovazione, la crescita delle imprese e quindi, in ultima istanza, un'occupazione di qualità. Parlo non solo come senatore, ma anche come imprenditore che lavora da decenni nel settore, con una profonda conoscenza dei meandri e delle sfide che le imprese italiane affrontano ogni giorno. Per capire la portata di ciò che abbiamo di fronte, dobbiamo comprendere qual è oggi la situazione in cui ci troviamo. Nonostante l'aumento delle risorse per gli incentivi avvenuto negli ultimi anni, la diffusione frammentata delle informazioni, la complessità delle procedure burocratiche, l'incertezza sull'erogazioni portano a una distribuzione inefficace delle risorse pubbliche e alla nascita di un mercato delle agevolazioni in cui gran parte delle risorse non ottengono il loro scopo primario, ma si disperdono nella lunga trafila burocratica. In Italia, migliaia di imprese ogni anno tentano di accedere agli incentivi che lo Stato mette a disposizione; sono risorse preziose, spesso fondamentali per poter innovare, assumere, formare. Ma il cammino per accedere a queste risorse è costellato di ostacoli. La burocrazia, la mancanza di chiarezza e la complessità sono nemici quotidiani delle nostre imprese. in discussione parte da presupposti corretti, a partire dai principi chiave, tra cui la stabilità delle misure, la misurabilità dell'impatto economico, la semplificazione delle procedure. Come Partito Democratico condividiamo in particolare la creazione di un codice degli incentivi per armonizzarne la disciplina; l'obiettivo di razionalizzare l'offerta di incentivi, evitando sovrapposizione e frammentazione del sostegno pubblico alle imprese; le misure per un miglior coordinamento tra gli incentivi statali e regionali, al fine di evitare duplicazioni e favorire la complementarietà tra le politiche regionali nazionali; la semplificazione dei controlli sulle attività economiche per migliorare l'efficienza e ridurre la burocrazia; le misure per la digitalizzazione e la trasparenza degli incentivi, con l'implementazione di strumenti come il registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma "incentivi.gov.it". Esprimiamo anche noi un forte apprezzamento per i lavori svolti in Commissione, sia per la gestione del Presidente che ha permesso un grande livello di approfondimento dell'esame in sede referente, sia per le aperture dimostrate dal Governo e dal relatore. Siamo in particolare soddisfatti che siano stati accolti positivamente emendamenti del Partito Democratico che hanno introdotto il principio della strategicità dell'interesse nazionale; l'obiettivo di favorire l'occupazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori e il coinvolgimento delle associazioni di categorie; di una richiesta che abbiamo avanzato non solo per l'efficienza del processo ma anche e soprattutto per ridare credibilità al rapporto Stato-cittadino, ovvero il divieto per la pubblica amministrazione di richiedere documenti e informazioni già in suo possesso. Il testo uscito dalla Commissione è frutto di un buon lavoro di analisi e di compromesso alto, e rappresenta un significativo passo in avanti rispetto al testo originale. La Commissione ha quindi dimostrato che un approccio collaborativo produce risultati concreti. Tuttavia, siamo convinti che possiamo e dobbiamo fare di più per le nostre imprese e per il tessuto economico del nostro Paese. Fra le varie proposte che non sono state recepite e che riteniamo fondamentali, ne elenco tre, perché danno la direzione e il senso del modello di sviluppo che il Partito Democratico vorrebbe per il nostro Paese: un'Italia più trasparente, più giusta, più ambientalmente sostenibile. Abbiamo chiesto e chiediamo di nuovo in quest'Aula che gli incentivi siano orientati al conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, superando i sussidi ambientalmente dannosi in favore di incentivi ambientalmente favorevoli. Abbiamo chiesto e chiediamo nuovamente in quest'Aula che vi sia un portale davvero unico nazionale, che raccolga in maniera trasparente qualsiasi tipo di incentivo pubblico, nessuno escluso, per porre davvero fine al mercato dell'intermediazione e permettere l'accesso a tutte le imprese, comprese quelle più piccole e meno strutturate. Abbiamo chiesto, e chiediamo di nuovo in quest'Aula, che venga inserita, come requisito premiante, la certificazione della parità di genere. Il nostro Paese, infatti, non riuscirà mai a esprimere tutto il suo potenziale fino a quando non ci sarà una parità reale di occupazione, di ruoli e di stipendi. Alcuni potrebbero obiettare che abbiamo già fatto abbastanza e che il provvedimento è già un passo avanti. Capisco questa posizione, ma permettetemi di dissentire. Quando ascolto le testimonianze dei miei colleghi imprenditori, io sento una richiesta unanime: servono più semplicità, più chiarezza, più modernità. Non possiamo fermarci ora. Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo l'opportunità di fare una vera differenza e dobbiamo coglierla. Concludendo, quello che chiedo a tutti noi oggi è non di ribaltare il disegno di legge, ma di affrontare l'esame in Assemblea con lo stesso spirito costruttivo avuto in Commissione. Dobbiamo pensare a quelle piccole imprese fatte di donne e uomini della nuova generazione, che magari da un *garage* o da un piccolo ufficio stanno cercando di crescere, di innovarsi, di dare lavoro. Questo provvedimento può essere uno strumento potente per loro e spetta a noi renderlo il migliore possibile.

io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi che si sono susseguiti. Devo dire che, in merito a questo disegno di legge n. 571, c'è veramente un un grande spirito di collaborazione: una collaborazione fattiva, volta perseguire degli obiettivi importanti per le nostre imprese. Questo perché l'impresa italiana è fulcro non solo della nostra economia

per un bel po' di tempo, ma noi ci troviamo di fronte anche alle difficoltà dettate dall'aumento dei tassi della BCE. E poi sappiamo quanto avvenuto con l'aumento del costo dell'energia e delle materie prime. Sono difficoltà

il senatore Russo - per citarlo per ultimo - serve la massima attenzione della politica e delle istituzioni. Condivido ciò, ma credo che questo provvedimento sia la dimostrazione di tale auspicio. Qui c'è stata veramente la massima attenzione da parte della politica e delle istituzioni. Pertanto, il sistema di revisione degli incentivi alle imprese, ma anche - come più volte è stato ribadito - le disposizioni di semplificazione delle relative procedure sono importanti, perché questo provvedimento è un collegato a quella che è la manovra di bilancio 2023-2025, in coerenza con le disposizioni previste Quindi, utilizziamo al meglio quelli che sono i fondi del PNRR e contrastiamo tutte le difficoltà con le quali le imprese sono chiamate chiamate ogni giorno a fare i conti. Questo ci proietta anche, con orgoglio, in un contesto internazionale dove il *made in Italy* è sempre più apprezzato e dove noi, anche attraverso questo

provenienti da mercati esteri che non prestano di certo attenzione nei confronti del mondo del lavoro o dello sfruttamento della manodopera minorile. Da noi, invece,

2.000 tipologie di incentivi, un terzo dei quali sono di carattere nazionale e due terzi di carattere regionale. C'è quindi bisogno di semplificazione

che non funzionano. Noi continuiamo a dire che le risorse ci sono. Il problema è che, se si hanno 2.000 tipologie di incentivi, questi sono troppo frastagliati per cercare di andare al punto. E siccome ce n'è bisogno, in questo momento particolare e in questo periodo storico (abbiamo avuto notizia in queste ore dei dati ulteriori e delle previsioni sul prodotto interno lordo), è chiaro che le risorse che sono a disposizione delle imprese per un rimbalzo dell'economia devono essere assolutamente puntuali. Concludo questo mio breve intervento ringraziando ancora e ricordando ricordando che questo *modus operandi* sta portando a un testo assolutamente migliore rispetto a quello di partenza. *(Applausi)*.

Colleghi, nessuno ha chiesto la votazione elettronica; di solito siete voi del MoVimento 5 Stelle che la chiedete.

Benvenuti in Senato.

Mi riferisco alle aree di crisi industriale complessa e alle aree che hanno un alto tasso di disoccupazione. Credevo che ci fosse la possibilità di un'intesa con la maggioranza verso un obiettivo comune, che è quello di

L'Italia, purtroppo, è caratterizzata da grandi divari territoriali: come pensate di risolverli, con l'autonomia differenziata? abbiamo avuto una vera e propria doccia fredda in Commissione, perché, proprio quando parlavamo dell'autonomia differenziata, abbiamo saputo della bocciatura da bilancio degli emendamenti che prevedevano una perequazione infrastrutturale tra le varie Regioni. Ciò significa che nelle intenzioni di questo Governo ogni Regione deve restare con ciò che ha acquisito finora, che gli investimenti infrastrutturali sono stati fatti magari nella Regione A e nella Regione B e tutte le altre devono andare avanti con le carenze infrastrutturali che ne impediscono la crescita. crescita. Il Sottosegretario ha fatto prima riferimento agli incentivi che non funzionano. Faccio un esempio: vivo nel territorio del piceno, dove c'è un'area industriale che è stata costruita con un incentivo che non ha funzionato o, meglio, ha funzionato finché era in essere, perché non c'era un progetto industriale organico alla base e perché sono stati incentivati investimenti produttivi non solo senza un disegno industriale organico, ma anche senza creare la complementarietà tra le imprese. Non sono stati fatti investimenti infrastrutturali e quindi, cessato l'incentivo, le aziende se la sono data a gambe. Questa è la realtà italiana. La cosa che però mi sorprende è che dovremmo anche cercare di vedere il contesto in cui viviamo in Europa. Le politiche europee sono tutte quante mirate a ridurre i divari tra le varie regioni europee,

allora di dare un indirizzo affinché gli incentivi vengano fatti laddove servono realmente significa anche stare al passo con quello che fanno i Paesi europei.

riformulazione. Guardiamo quello che stanno facendo intorno a noi: anche gli stessi fondi strutturali europei hanno la finalità di ridurre i divari territoriali. Non è possibile che in un provvedimento come quello al nostro esame non si trovi spazio per una finalità strategica.

Capisco benissimo l'intervento, ma i temi legati alla coesione territoriale sono già inseriti nei principi della delega

Giuliano Montaldo, cineasta e intellettuale tra i più significativi del nostro Paese. Montaldo è scomparso lo scorso 6 settembre, proprio nei giorni dello svolgimento della Mostra del Cinema di Venezia, dove aveva esordito, poco più che trentenne, nel 1961. Ed a Venezia resterà per sempre legato, per avere molti anni dopo, negli anni Ottanta, girato quel "Marco Polo" che, a tutt'oggi, è la serie italiana più venduta alle televisioni di tutto il mondo. Montaldo è stato autore di grande talento e poliedricità e di grande spessore. In particolare, non smise mai il tratto di un cinema dal fortissimo impegno civile. I suoi film sono atti d'accusa rigorosi contro la degenerazione del potere, contro l'intolleranza e le discriminazioni, contro le ingiustizie. "Sacco e Vanzetti", la sua pellicola ebbe un grande successo internazionale e fece conoscere all'opinione pubblica italiana la storia di due lavoratori innocenti, che, negli Stati Uniti in preda all'ossessione anticomunista, vennero ingiustamente uccisi, per la colpa di essere anarchici, per la colpa di essere poveri, per la colpa di essere italiani e per la colpa di essere stranieri in terra straniera. E fu grazie a quel film che accadde un atto politico di enorme rilievo: la completa riabilitazione, da parte dello Stato del Massachusetts, dei nostri due connazionali. Montaldo, con il suo lavoro, contribuì potentemente alla costruzione di una coscienza storica. Penso al suo "Giordano Bruno", anch'esso interpretato da Gian Maria Volonté, e a "L'Agnese va a morire", il primo lavoro cinematografico sulla Resistenza con una donna protagonista: un ritorno al Neorealismo, contro il rischio del revisionismo storico che Montaldo vedeva; la bicicletta di Agnese, staffetta partigiana uccisa dalle SS, a rappresentare il romanzo popolare ed epico, che è a fondamento della nostra Repubblica. Giuliano Montaldo, giovanissimo, scelse di appartenere a quella nuova Italia. Fu partigiano e, dopo la Resistenza, da Genova arrivò a Roma, dove visse con Elio Petri e Gillo Pontecorvo, di cui fu assistente nella realizzazione de "La battaglia di Algeri". Fu uno dei protagonisti della grande stagione del nostro cinema. «Non sappiamo imparare dalla storia», disse dopo lo scoppio della guerra di aggressione contro l'Ucraina. Ed il valore della memoria è traccia costante del suo lavoro lungo l'arco, durato quasi un secolo, della sua esistenza, vissuta sempre al fianco del grande amore della sua vita, Vera Pescarolo. Montaldo aveva la capacità rara e l'intelligenza di parlare ai più giovani, da insegnante del Centro Sperimentale di Cinematografia, da e da attore, la sua passione, come nell'ultimo suo personaggio: un indimenticabile poeta novantenne che insegna al ragazzo disilluso che lo accompagna ad accorgersi della vita e a riempirla di passione e di bellezza, rispettando gli altri e, in questo, ritrovando se stessi. *(Applausi)*.

colpi di pistola, sparati all'impazzata nella notte, hanno gelato il sangue degli abitanti di un quartiere balzato tragicamente alla ribalta delle cronache per le reiterate violenze subite da due cuginette. Le parole pronunciate da don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, rendono l'idea del clima teso che si respira in quel territorio: «Per la gente della mia parrocchia non c'è pace», scrive su Facebook. «In sella «In sella alle loro moto sono arrivati ancora una volta. Volti coperti, armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando all'impazzata. È il terrore. Le "stese" fanno paura. Può morire chiunque. Signore, aiutaci». Se ne avete il coraggio, venite voi con i vostri figli ad abitare al Parco Verde di Caivano. Forza, fratelli e sorelle onesti del Parco Verde, coraggio: il Signore non ci abbandona. Di nuovo ieri mattina l'antistato è tornato a ruggire prepotentemente, sparando ancora in via Pio IX contro un'auto parcheggiata in strada, con l'obiettivo chiarissimo di rimarcare il proprio predominio su un territorio già martoriato. E se in quell'auto si fossero trovate delle persone, magari dei bambini, come accadde a Silvia Ruotolo, Annalisa Durante o Genny Cesarano, freddati da proiettili vaganti nel corso di sparatorie? Ben venga il controllo del territorio, purché non episodico, ma strutturale. Non ho nulla contro l'operazione interforze deliberata dal Governo per far sentire la presenza dello Stato, ma mi chiedo: quale Stato?

L'articolo 3 della nostra Costituzione afferma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Torno a ribadire a distanza di una settimana che non basta mostrare i propri muscoli: la vera rivoluzione dev'essere culturale e sociale e deve ripartire in primo luogo dalla scuola, che invece è sempre più liquefatta e depotenziata. Onorevoli colleghi e colleghe, negli ultimi giorni questo Esecutivo ha deciso di alzare la propria voce solo perché il dibattito pubblico e i *mass media* hanno costretto l'agenda politica a inserire all'ordine del giorno la parola «Caivano»;

Esiste una Caivano in ogni Comune in cui non vengono garantiti i livelli essenziali delle prestazioni, disciplinati dall'articolo 117 della Costituzione e mai definiti; esiste dove lo Stato non ha erogato nemmeno un centesimo per i propri asili nido, com'è avvenuto ad Altamura e in tantissime altre realtà del Meridione; esiste nei Comuni che, con il definanziamento del PNRR, subiranno un taglio di svariati miliardi di euro, e ancora, nei Comuni del Centro-Sud a cui non verranno riconosciute opere per 2,5 miliardi di euro, così come voluto dal ministro Salvini. Non servono decreti che portino il nome di un singolo Comune, non servono passerelle; abbiamo bisogno di uno Stato che ritorni nei territori che ha preferito abbandonare. Abbiamo bisogno di risposte ora e subito.*(Applausi)*.